colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato il calendario dei lavori fino al 22 settembre. Rimane confermata per la seduta pomeridiana di oggi la discussione dei disegni di legge recanti rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato. In apertura della seduta pomeridiana di martedì 20 settembre, sarà commemorata la figura di Mino Martinazzoli. I Gruppi potranno intervenire per 10 minuti ciascuno. Seguirà un'informativa del Governo sull'incidente avvenuto in una fabbrica di Arpino. Nella seduta antimeridiana di mercoledì 21, il Ministro della giustizia renderà comunicazioni all'Assemblea sul sistema carcerario e sui problemi della giustizia. Data 1'importanza del tema, il dibattito conseguente impegnerà anche la seduta pomeridiana di mercoledì. Il calendario dei Il calendario dei lavori della prossima settimana prevede inoltre 1'esame del disegno di legge in materia di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, ratifiche di accordi internazionali e documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. La Conferenza dei Capigruppo ha altresì stabilito la calendarizzazione per il pomeriggio di martedì 27 settembre della mozione Finocchiaro sull'istituzione di una Commissione speciale per l'esame di proposte di riforma costituzionale. È stata infine richiesta la disponibilità del Governo a rendere un'informativa sulla chiusura dello stabilimento FIAT di Valle Ufita (Avellino).

nuova finestra") ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011***

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'impostazione del provvedimento conferma la messa a regime nel 2010 del nuovo impianto di classificazione del bilancio per missioni e programmi, già adottato nel biennio 2007-2008, fatto proprio dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, al fine di assicurare una maggiore aderenza nella rappresentazione degli utilizzi delle risorse disponibili rispetto alle finalità e ai risultati dell'azione di governo. In relazione alle risultanze registrate nel 2010 dal rendiconto generale dello Stato, va segnalato che il disegno di legge evidenzia un avanzo di competenza, per le operazioni complessive, in crescita rispetto al 2009. Esso mostra però, per le sole partite finali, un disavanzo di competenza (un dato comunque molto migliore del disavanzo del 2009, allorché si era registrato già un miglioramento rispetto al dato 2008). Sul versante della spesa, il risultato di competenza ha risentito in senso attenuativo del risultato complessivo conseguito dalle economie di gestione. Nel medesimo senso, anche il saldo di cassa riferito alle operazioni finali, che conferma per il 2010 un risultato di segno negativo, dato tuttavia che si presenta in leggero miglioramento a fronte del 2009. Gli andamenti registrati nel 2010 evidenziano poi un miglioramento per il saldo delle partite finali, che hanno portato a segnalare un indebitamento netto di competenza pari a meno 17.900 milioni di euro

Tale dato, sul versante della cassa, ha registrato una diminuzione del divario negativo delle entrate rispetto alle spese. È da segnalare come significativo elemento di novità, in senso senz'altro positivo, anche un incremento della misura del risparmio pubblico di competenza, che si attesta nel 2010 a più 28.742 milioni di euro (cioè l'l,9 per Il medesimo risparmio pubblico, espresso invece in termini di cassa, evidenzia un sensibile miglioramento, essendosi attestato a meno 10.154 milioni di euro, a fronte del dato 2009 che era stato di meno 15.984 milioni di euro. In termini di competenza, il 2010 ha registrato anche un lieve incremento del ricorso al mercato, che si attesta al 13,6 per Un'analoga tendenza in rialzo si registra anche per il ricorso al mercato espresso invece in termini di cassa, che si attesta nel 2010, sempre in valore assoluto, a 248.950 milioni di euro (cioè il 16,1 per cento del PIL), a fronte dei 243.148 milioni registrati nel 2009. Nel 2010 si conferma nella sostanza anche una notevole differenza tra ricorso al mercato, in termini di competenza, e l'analogo valore del titolo IV delle entrate. La differenza è - come noto - da imputare agli effetti della gestione del bilancio. In particolare, poi, sul versante della cassa, l'esercizio 2010 ha registrato incassi per operazioni finali ammontanti a 444.142 milioni di euro, pari al 99,25 per cento delle previsioni definitive. In merito alla dinamica degli incassi, si segnalano poi, in particolare, le risultanze in sensibile decremento del gettito tributario 2010 che per il titolo I si attestano su di un valore pari a 408.952 milioni di euro. Tale dato rappresenta il 92 per cento degli incassi finali complessivi del 2010. Sempre per i profili di cassa, è poi da sottolineare anche il sensibile decremento registrato, in valore assoluto, nel gettito delle entrate extratributarie (titolo II) rispetto al gettito del 2009, a cui si affianca l'analogo andamento negativo segnato dalle entrate per alienazione di beni patrimoniali del titolo III, dopo la buona *performance* registrata nel 2009. Dal lato della spesa, il 2010 ha registrato pagamenti per operazioni finali al lordo delle regolazioni debitorie pari a 503.988 milioni di euro, equivalenti all'88,8 per cento delle corrispondenti autorizzazioni. Dell'ammontare complessivo dei pagamenti finali, 452.441 milioni di euro sono riferibili a spese di parte corrente, mentre 51.547 milioni di euro sono riconducibili a spese in conto capitale. Quindi abbiamo praticamente il 10 per cento e il 90 per cento del valore che ho letto poc'anzi. Il ritmo di realizzazione delle spese si è dunque attestato nel 2010 -considerando anche i residui di nuova formazione - su di una percentuale complessiva analoga a quella segnata nei precedenti esercizi e pari all'87,4 per cento confermando un elevato livello di velocità delle procedure di erogazione già evidenziatosi nei consuntivi degli ultimi anni. sottolineare due aspetti che sono stati oggetto della discussione in Commissione da parte dei colleghi. Mi riferisco ad argomenti trattati anche in precedenti discussioni di rendiconto relativamente ai residui passivi e attivi e in particolare sui passivi e sulla loro gestione

Signor Presidente, l'articolo 33 della legge di contabilità stabilisce che entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre. Sulla base del comma 3 del medesimo articolo 33, con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione, ivi comprese le spese predeterminate predeterminate per legge, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Venendo ai dati contenuti nel disegno di legge di assestamento per il 2011, si evidenzia anzitutto un miglioramento dei saldi di bilancio in termini di competenza, Grazie, infatti da 40.640 milioni a 32.107 milioni, con un miglioramento di 8.534 milioni di euro, pari a circa il 21 per cento rispetto all'entità del medesimo aggregato indicata dalla legge di bilancio; detto importo deriva dalla somma algebrica tra un peggioramento di 1.350 milioni, dovuto a variazioni per atto amministrativo, e un miglioramento per 9.884 milioni derivante dalle proposte dell'assestamento stesso. Tali variazioni derivano in particolare dalla riduzione delle spese per rimborso prestiti, in misura di 16.254 milioni, ivi compresi gli atti amministrativi; la relazione al disegno di legge in esame chiarisce che la proposta riduzione di 16 miliardi è riferita per 10 miliardi alle minori necessità di concambi tra i nuovi CCT euro e i vecchi CCT e per 6 miliardi a un uso inferiore, rispetto a quello previsto inizialmente, dello strumento delle *commercial paper.* paper.* Le entrate finali - per effetto delle variazioni per atti amministrativi e delle variazioni proposte con il presente provvedimento - aumentano, in termini di competenza, di 8.618 milioni rispetto alle previsioni iniziali. La variazione positiva riconducibile al presente provvedimento è pari a 7.689 milioni, mentre l'incremento positivo associato alle variazioni per atti amministrativi è pari a complessivi 929 milioni. In sostanza, signor Presidente, questo passaggio sottolinea come le manovre messe messe in campo dal Governo negli ultimi anni abbiano avuto un'effettiva credibilità ed attuazione, ed evidenzia una tenuta sull'assestamento 2010. La variazione delle entrate tributarie riguarda sia le imposte dirette sia quelle indirette. In particolare si registra una riduzione dell'IRE per 1.592 milioni e un aumento dell'IRES per 3.727 milioni. Inoltre, diminuiscono le entrate derivanti dall'imposta sostitutiva e dalle ritenute di acconto sugli utili delle persone giuridiche nella misura, rispettivamente, di 1.751 milioni e 173 milioni. Per quanto riguarda l'IVA, invece, si evidenzia un incremento di 5.162 milioni rispetto al previsionale. La relazione illustrativa del provvedimento indica come voci di maggior gettito anche quelle relative alla imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastale sui contratti di locazione immobiliare (in misura di 1.087 milioni) e alla cedolare secca sui contratti di locazione (in misura di 2.751 milioni). In proposito, si rammenta che a decorrere dal 2011, in base all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, è prevista la facoltà di applicare una cedolare secca sul canone di locazione annuo sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché dell'imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione. In merito a questo, in Commissione c'è stato un dibattito in cui il Governo ha dato chiarimenti rispetto alla compensazione, essendo questa una facoltà del contribuente, tra il gettito della cedolare secca e l'eventuale diminuzione dell'IRE. Per quanto riguarda invece l'imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastale sui contratti di locazione immobiliare, si ricorda che essa è stata introdotta dall'articolo 1, comma 16, della legge di stabilità per il 2011, che determina l'obbligo per le parti di versarla in unica soluzione entro il 31 marzo 2011. Nel complesso, si segnala che, anche per l'esercizio finanziario 2011, l'aggiornamento puntuale del gettito non risulta possibile al momento della presentazione alle Camere del disegno di legge di assestamento, a causa della mancanza dei dati completi concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi. Passando all'assestamento delle previsioni in termini di cassa, queste determinano nel 2011 un peggioramento dei saldi. Le variazioni disposte per atti amministrativi hanno infatti incrementato la spesa di 1.979 milioni, mentre le proposte dell'assestamento incrementano le autorizzazioni delle spese finali per 9.355 milioni; le spese finali aumentano quindi di 11.334 milioni. Per quanto riguarda le entrate, esse aumentano in misura di 8.648 milioni. Nel complesso l'aumento del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA, è quindi pari a 2.689 milioni di euro. Nello specifico, la differenza è riconducibile al lato della spesa, nel quale si registra un incremento delle dotazioni di cassa per 11.334 milioni, laddove in termini di competenza la variazione delle corrispondenti voci risulta nell'aggregato trascurabile (85 milioni). L'aumento delle dotazioni di cassa deriva da incrementi per 9.385 milioni della spesa primaria corrente e per 7.830 milioni delle spese in conto capitale, solo in parte controbilanciati dalla diminuzione della spesa per interessi di 5.888 milioni. I trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche rappresentano una voce in relazione alla quale le variazioni sono sensibilmente più elevate in termini di cassa che di competenza: si tratta infatti di un aumento di 10.334 milioni a fronte di 4.033 milioni. La relazione illustrativa evidenzia che 5.120 milioni di euro, cioè una gran parte di questo scostamento, sono in relazione ai trasferimenti agli enti di previdenza e assistenza. in Commissione ha spiegato che si tratta dello scostamento degli impegni del Ministero rispetto agli impegni soprattutto dell'INPS. Per quanto riguarda invece la spesa in conto capitale, gli incrementi più consistenti delle dotazioni di cassa (in valore assoluto e nel confronto con le corrispondenti variazioni in termini di competenza) riguardano i contributi alle imprese. Quanto alla gestione in conto residui, va segnalato che al 31 dicembre 2010 i residui passivi accertati per le spese finali di bilancio statale, al netto di quelli relativi al rimborso dei prestiti (pari dei prestiti (pari a 74 milioni), ammontavano a 108.203 milioni, dei quali 66.686 milioni derivano dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2010. A fronte di un dato complessivo dei residui 2009 pari a 95.926 milioni per le spese finali, l'aumento è imputabile esclusivamente alla parte corrente, che registra un incremento da 50.059 milioni a 65.621 milioni. I residui in conto capitale scendono invece da 45.867 a 42.582 milioni. Nell'ambito dell'incremento di 15.562 milioni dei residui correnti, le voci più significative sono costituite dai trasferimenti agli enti previdenziali, che aumentano di 9.148 milioni e da quelli alle Regioni, che aumentano di 8.079 milioni. La relazione illustrativa al disegno di legge in esame segnala che, nell'ambito di tale ultimo importo, 6.961 milioni riguardano le erogazioni alle Regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA derivante dall'accantonamento della quota premiale del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda lo scostamento dei residui accertati rispetto ai residui presunti, si rileva che l'unico anno in cui i residui accertati sono stati inferiori a quelli presunti è stato il 2002; tale effetto potrebbe essere

Si evidenzia che, dopo la rilevante contrazione dello scostamento tra la consistenza presunta e quella effettiva dei residui passivi verificatasi con riferimento all'anno 2007, il *trend* ha ripreso a salire nel 2009, raggiungendo il 112,1 per cento Infine, l'articolo 2 del provvedimento reca alcune modifiche all'articolo 2 della legge di bilancio per il 2011, a partire da quella indicata al comma 1, lettera *a)*, dove si propone l'aumento del limite massimo di emissione di titoli pubblici a 75 miliardi. Si ricorda, in proposito, che generalmente la legge di assestamento provvede a ridefinire in aumento il limite di emissione, registrando le modifiche degli obiettivi di fabbisogno intervenute o previste nel corso dell'esercizio. A partire dall'esercizio 1991, il limite massimo dell'emissione dei titoli è stato quasi sempre fissato ad un livello in linea con le previsioni del fabbisogno, realizzando in tal modo una sorta di margine di sicurezza. Quanto alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, ivi si interviene sull'articolo 2, comma 7, della legge di bilancio per il 2011, nella parte in cui viene fissato l'importo del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge n. 196 del 2009; tale importo viene innalzato a 12.000 milioni. In proposito, nel rilevare che le variazioni al bilancio per atti amministrativi già registrano un aumento delle autorizzazioni di cassa pari a 7.235 milioni, si sottolinea che l'indicato innalzamento del limite di importo del fondo cassa, come già evidenziato nella precedente trattazione relativa ai prelievi dai fondi di riserva, sembrerebbe suggerire una limitata attendibilità delle previsioni iniziali relative alle dotazioni di cassa. Quanto alla modifica della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2 ivi si dispone poi che all'articolo 2 della legge di bilancio per il 2011 venga aggiunto un nuovo comma, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra gli stanziamenti dei capitoli n. 2751 e 2752 dello stato di previsione del proprio Ministero per l'anno finanziario 2011. I due capitoli indicati sono relativi a somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, con riferimento a IVA e dazi. In Commissione, signor Presidente, sono stati approvati tre emendamenti del Governo, il primo dei quali - 1.Tab.3.1 - si riferisce sostanzialmente

nonché le spese per costruzione e acquisizione di impianti, eccetera alle effettive esigenze, tenuto conto dell'adempimento degli impegni internazionali e degli aggiornamenti del programma di investimenti strategici di elevata priorità. nella sostanza il più importante (2 miliardi e 400 milioni di euro), approvato dalla Commissione, riguarda il dettaglio in norma degli accantonamenti della legge di stabilità per la salvaguardia sul provvedimento di entrate legato all'asta delle frequenze radiotelevisive. Tale accantonamento

sarebbero andati a beneficio dei saldi di finanza pubblica anche se si fossero verificate quelle entrate previste per l'asta famosa, come poi tra l'altro si sta verificando. Anzi, si parla di entrate sovrabbondanti rispetto alla previsione di 2 miliardi e 400 milioni, ma tali tagli sono resi effettivi dalla norma di assestamento a beneficio dei saldi di finanza pubblica. Sostanzialmente vanno a rafforzare le manovre messe in campo nel corso dell'anno 2011.

*(PD)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, mi soffermerò in modo particolare sul rendiconto, ritenendo che sia essenziale recuperare, nell'analisi dell'intero ciclo di bilancio, una maggiore attenzione sui risultati dell'esercizio. discutendo - e penso che sia un fatto positivo - sulla modifica dell'articolo 81 della Costituzione. Proprio l'esigenza di questa modifica ci richiama al fatto che le cautele poste nel processo *ex ante*, che sono ben individuate nell'articolo 81 della Costituzione, non sono state sufficienti alla formazione di un debito così elevato. Ci richiama pure al fatto che il rispetto formale dell'articolo 81 sia però stato accompagnato, nella lunga storia della Repubblica, anche da violazioni sistematiche della sostanza. Quindi, dobbiamo assolutamente centrare centrare la nostra attenzione sul fatto che ci sono insufficienti elementi conoscitivi *ex post* che condizionano l'efficacia e i risultati della spesa pubblica. Pertanto è molto importante che si proceda alla modifica dell'articolo 81 della Costituzione non tanto, come impropriamente si afferma, sul principio del pareggio di bilancio, quanto piuttosto sul principio della sua sostenibilità. non è affatto la rinuncia ad usare lo strumento del bilancio pubblico come strumento di politica economica, ma l'affermazione che solo un bilancio sano, sano, non stressato da squilibri strutturali, consente di porre in campo politiche pubbliche attive, tese a promuovere la crescita e a rimuovere i fattori di eccessiva diseguaglianza. Dovremo anche dare un giudizio politico sul fatto che i bilanci pubblici escono stressati da questa fase di grande crisi crisi globale della finanza; sono stressati - volendo usare un termine un po' forte - dall'avidità privata, perché la grande crisi dei bilanci pubblici nasce negli Stati Uniti da un eccesso di diseguaglianza che ha fatto promuovere strumenti di finanziamento dell'investimento delle famiglie più povere. Questo eccesso di finanziarizzazione ha portato a fallimenti privati che sono stati risanati da risorse pubbliche, i bilanci pubblici appesantiti dai fallimenti privati ora richiedono costi di servizio del debito più elevati di prima: quindi, un enorme spostamento di risorse da politiche pubbliche al risanamento di fallimenti privati. solo un bilancio sano può consentire di sviluppare le necessarie politiche economiche positive per la crescita e l'eliminazione delle diseguaglianze.

un chiaro *commitment,* coerente e condiviso, in merito alla necessità di gestire i bilanci in modo sostenibile, di una conseguente modifica delle leggi di contabilità e degli stessi Regolamenti parlamentari, di un attento monitoraggio della spesa e di un'accurata*spending* *review*. Approfitto dell'occasione per dire che naturalmente tutte queste considerazioni portano al fatto che dovremmo dare attuazione a quell'iniziativa volta alla creazione di un Servizio unificato del bilancio di Camera e Senato, più volte proposta e mai attuata. Ho fatto questa premessa perché i risultati del bilancio consuntivo quest'anno ci dicono delle cose importanti che è bene sottolineare. Intanto c'è un risultato che non va sottovalutato. Per la prima volta la spesa corrente,

il ritardo con cui il Governo ha percepito questa necessità, perché per tutto il 2008 e anche fortemente. Quindi, con un ritardo di due anni si è percepita la necessità di arrivare a procedure di contenimento della spesa. bisogna guardare anche la qualità della spesa, perché la spesa va contenuta ma ne va migliorata anche la qualità e qui emergono dei dati preoccupanti. Abbiamo una riduzione del 25,2 per cento dei consumi intermedi, risultato molto importante, ma bisognerà capire quanta parte di questa riduzione avrà un rimbalzo nell'esercizio in corso, perché come vediamo dall'affannoso inizio dell'anno scolastico si possono anche ottenere dei risparmi considerevoli ma a prezzo di mettere in discussione il buon funzionamento dei servizi. Abbiamo una riduzione del 32,6 per cento dei trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali: sono 2 miliardi di euro in meno sottratti al sostegno dei redditi più deboli e quindi non dobbiamo meravigliarci se ciò ha effetto sulla riduzione dei consumi. Abbiamo una riduzione complessiva delle spese in conto capitale

che ci portano a constatare che a luglio 2011, rispetto al luglio 2010, c'è stata una crescita del debito per il complesso delle amministrazioni pubbliche del 3,9 per cento, cifra in sé considerevole

c'è un crescita molto più veloce del debito dello Stato centrale rispetto a quanto avvenga per lo Stato periferico. Viceversa le manovre di contenimento della spesa che il Governo ha predisposto pesano di più sul comparto locale, che è quello che ha messo in atto comportamenti più virtuosi. Infine, avviandomi alla conclusione, osservo che la Corte dei conti nel suo giudizio di parificazione mette in luce alcuni aspetti problematici di gestione che è bene che il Governo si impegni a migliorare. Ad esempio, c'è un utilizzo di capitoli promiscui, senza distinzione di spese per consumi, per personale, per trasferimenti, e ciò rende meno efficace il giudizio sulla trasparenza del bilancio. C'è un utilizzo diretto di fondi costituiti in bilancio senza che vengano attribuiti agli ordinari capitoli di spesa al momento degli impegni, determinando perciò problemi di classificazione e di rispetto, ancora una volta, dei criteri di trasparenza e leggibilità del bilancio. Non c'è un rispetto pieno delle norme di trasparenza e imparzialità per i lavori, sia pure di minore importo; c'è quindi un lavoro di miglioramento importante da fare. Concludo dicendo che tutto ciò sottolinea l'importanza di attuare sul serio quell'impegno ad una generale *spending review* della spesa pubblica che, per iniziativa dell'opposizione, e del PD in particolare, è stata inserita nell'ultima manovra finanziaria. Il consuntivo del 2011 non ci consentirà di avere già gli effetti di questa revisione. Mi auguro, però, che la sua discussione avverrà in un contesto in cui vedremo pienamente attuato questo importante processo di revisione della spesa pubblica.

ringrazio lei e i colleghi, dopo l'apertura di questa discussione generale ad opera dei due relatori, per la qualità degli interventi che si stanno producendo nell'analisi di un provvedimento come questo. L'analisi del rendiconto relativo all'esercizio 2010 rende infatti evidente l'impegno di questo Governo e di questa maggioranza per quella fermezza contabile che è precondizione per il risanamento dei conti pubblici, a sua volta precondizione per qualsiasi opera opera di sviluppo che si voglia intraprendere. Basti vedere i saldi, quei rapporti che sinteticamente evidenziano l'andamento delle componenti attive e passive dei bilanci pubblici. Ebbene, dal risparmio pubblico al ricorso al mercato, tali indicatori sono tutti in trasformazione positiva. Un andamento positivo che si registra già nell'aspetto previsionale. In effetti, a parte la sostanziale equivalenza nella variazione di entrate e spese complessive, in cui appare evidente la significativa riduzione delle entrate classificate come «accensione prestiti», ridottesi di oltre 32 miliardi, le previsioni definitive di competenza, relative alle entrate finali, fanno registrare un netto aumento di circa 4,5 miliardi ed uno, molto più contenuto, delle spese finali, per 1,5 miliardi. Importi che, se scomposti, poi, appaiono ancora più significativi. Per le entrate, infatti, è evidente la crescita di quelle correnti, per oltre 3,5 miliardi, nonostante la leggera contrazione di quelle tributarie; mentre dal lato delle spese, la cifra di 1,5 miliardi è data dalla somma algebrica dell'aumento di circa 7 miliardi di quelle in conto capitale e della riduzione di oltre 5 miliardi di quelle correnti. E qui non posso non segnalare che un significativo apporto è stato dato dai consumi intermedi, categoria di spesa nell'occhio del ciclone, più volte analizzata negli interventi in quest'Aula, la cui variazione evidenzia una diminuzione del 24 per cento rispetto al 2009. E questo a tutto vantaggio di un controllo di quella spesa dove, tra opacità e pieghe di bilancio, è sempre stato difficile contrarre i numeri. Queste sintetiche indicazioni comportano riflessi positivi dell'ordine di 9,5 miliardi, 3,3 miliardi, 6,8 miliardi e 36,9 miliardi rispettivamente per risparmio pubblico, saldo netto da finanziare, indebitamento netto e ricorso al mercato. E qui, signor Presidente, vorrei far presente che un grosso apporto al miglioramento di cui ho detto prima viene proprio dall'assestamento. Basti ricordare che sono a carico di questo provvedimento, solo come esempio, 8 dei 9,5 miliardi che costituiscono la differenza del risparmio pubblico a preventivo ed a consuntivo.

Gli accertamenti riferiti alle entrate correnti e finali sono in significativo aumento rispetto al dato delle previsioni definitive, e sostanzialmente in linea con i risultati del 2009 (la variazione, infatti, è solo dello 0,5 Gli impegni per le spese correnti e finali registrano invece una significativa riduzione, intorno ai 17 miliardi, che fa migliorare l'importo definitivo, sia rispetto a quello delle previsioni, che all'importo registrato lo scorso anno, la cui variazione è di meno 2,5 La gestione, quindi, apporta un significativo miglioramento ai saldi: una cifra che, in media, si aggira intorno ai 41,5 miliardi per risparmio pubblico, saldo netto da finanziare e indebitamento netto. 78, invece, i miliardi che impattano positivamente sul ricorso al mercato, soprattutto in un momento delicato e difficile come quello che stiamo vivendo; senza dimenticare la crescita di circa il 18 per cento rispetto al 2009 fatta registrare dell'avanzo primario pari a circa 48 miliardi, poco più del più del 3 per cento del PIL, un dato rilevante, anzi rilevantissimo, in considerazione dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico. A questo punto, signor Presidente, credo che sia opportuna una breve puntualizzazione, che forse potrebbe favorire una valutazione più spassionata dei reali andamenti della finanza pubblica. I saldi di cui stiamo parlando sono calcolati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili (in estrema sintesi, le partite contabili pregresse riferite ad entrate o spese che hanno già manifestato il loro impatto sull'economia). partite rilevanti, che vanno appunto "regolate", rappresentate in bilancio, che, ricordo, è ispirato a principi di chiarezza ed integrità. Solo per fare un esempio, l'indebitamento netto, il dato più sensibile per le valutazioni internazionali sulla finanza pubblica, in valore assoluto è pari a circa 66 miliardi nelle previsioni definite e a 59 miliardi nella gestione, importi che al netto di tali regolazioni diventano 54 miliardi per le previsioni e, addirittura, 13 per la gestione. L'andamento dei saldi, però, è la descrizione numerica di scelte operate da un Governo. In tal senso, quindi, essi testimoniano non solo l'impegno assicurato, ma anche le azioni intraprese da questo Governo e dalla maggioranza che lo sostiene, per mantenere gli impegni in materia di finanza pubblica concordati con i partner europei. Le risultanze contabili del rendiconto 2010, quindi, testimoniano, da un lato, le misure adottate a sostegno dell'economia: mi riferisco a quelle adottate anche negli anni immediatamente precedenti, come ad esempio le misure in favore di famiglie ed imprese oppure per ammortizzatori sociali, varate rispettivamente nel febbraio e nel luglio del 2009. Dall'altro lato, il rendiconto testimonia il mantenimento del rigore nei conti pubblici. Sono andate in questa direzione, infatti, quelle misure correttive degli andamenti, opportunamente mantenute per per il protrarsi della congiuntura negativa, di quella crisi nei mercati finanziari che in tempi più recenti ha significato l'attacco speculativo ai debiti sovrani, compreso quello del nostro Paese. Un bilancio in ordine, auspicabilmente in pareggio, è la migliore risposta che si può dare ai risparmiatori, ai cittadini italiani e ai mercati internazionali. Lasciamo quindi che parlino i numeri ed abbandoniamo sterili sterili speculazioni politiche, che in questo momento non aiutano il Paese ad affrontare e a vincere questa straordinaria sfida con i mercati internazionali.

si aggettiva duramente il bilancio dello Stato ed al quale faceva riferimento nei suoi discorsi il compianto presidente Cossiga, dicendo che è inutile guardare i bilanci, tanto sono tutti falsi.

in termini di comunicazione, una certa confusione. Infatti, quel che molto spesso è abbastanza falso è il documento che indirizza il bilancio, cioè la legge di stabilità oggi, anche se molto meno che nel passato, e la legge finanziaria in passato. questa, negli anni cui si riferiva il presidente Cossiga, spesso e volentieri, per giustificare delle uscite che erano ritenute necessarie dal voto parlamentare, quindi dalla politica, si finiva per sopravvalutare le entrate tributarie,

essere stimolato dalla loro attenzione rispetto alla nostra discussione che, essendo svincolata dalle altre discussioni che facciamo al momento in cui lavoriamo i documenti di bilancio e votiamo le manovre

realtà incontrovertibile dei numeri, come vanno le cose. Rispetto ad una critica politica che rileva

è abbastanza confortante, perché i numeri finiscono per far trasparire quel rigore che ormai sottolineo ormai, e lo dico con piacere, per aver partecipato tante volte ai lavori, alle puntualizzazioni e alle modifiche delle leggi di contabilità - sembra a questo punto assunto dai documenti di bilancio.

le spese per il rimborso dei prestiti, che non rappresentano una volontà ma l'evenienza nella trattazione dei titoli, sono l'unico elemento che varia le spese complessive. Con ciò voglio dire che nell'assestamento come nel rendiconto non manca certamente il rigore. Anzi, di rigore ce n'è stato parecchio e ciò si evidenzia in tutte le tabelle poste

di assestamento per ben due volte sono state negate, nel senso che viene rilevata una diminuzione dei fondi FAS già appostati nella legge di stabilità del 2011,

la risposta dei Ministeri interessati è intervenuta dopo il 31 maggio) si aggiungono altri spostamenti per 970 milioni di euro, che sono giustificati da provvedimenti legislativi che abbiamo approvato all'inizio dell'anno. Quindi, sull'unica partita di crescita contenuta nel bilancio, pari a circa 2 miliardi di fondi nazionali FAS, si registra uno storno totale; è questo ciò che mi preoccupa. Da un lato mi preoccupa e dall'altro mi conforta, sono stati questi appostamenti che hanno incoraggiato la nostra azione nell'approvazione dell'ultima manovra e che ci hanno consentito di chiedere il mantenimento dei fondi regionali, nella speranza che essi possano

la discussione sulla manovra di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziare 2011 ed il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziare 2010 arriva in Aula proprio nel giorno in cui l'ultimo bollettino di Bankitalia registra l'ennesima impennata del debito pubblico italiano, che è salito nuovamente a luglio scorso raggiungendo il livello *record* di 1.911,807 miliardi di euro, (ossia 10 miliardi di euro in più rispetto a giugno quando, per la prima volta, aveva superato la barriera dei 1.900 miliardi di euro) con un gravame di 31.863 euro a carico di ognuno dei 60 milioni di residenti, compresi i nascituri, i nascituri, e un fardello di quasi 87.000 euro su ogni famiglia. Il Governo, a parte le chiacchiere e le manovre seriali imposte dopo il commissariamento da parte della Banca centrale europea, non sta affrontando la riduzione del debito pubblico - questo è il problema - a cominciare dalla vendita di oro e riserve di Bankitalia, che non sono dei banchieri centrali ma del popolo italiano, con misure analoghe a quelle degli altri Paesi, anche per calmierare il prezzo dell'oro arrivato ad un livello *record*, che ostinatamente Trichet e Draghi continuano a difendere con le unghie e con i denti. Se non vi sarà un'inversione di tendenza, stabilendo

Signor Presidente, questo è un Paese che non cresce, con una produzione che continua a calare. Secondo gli ultimi dati dell'ISTAT

forniture di energia (3,8 per cento). Tale situazione è destinata ad aggravarsi perché i consumi stagnano,

Bisognerebbe cambiare paradigma e farsi sentire anche in Europa durante le riunioni dei Ministri economici e finanziari, e anche a livello di G20, quando si svolgono le riunioni cui partecipa il signor Ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, un economista come Paul Krugman - che, tra l'altro, è anche premio Nobel per l'economia - ha bacchettato

Krugman ha affermato testualmente: «I custodi miopi della stabilità dei prezzi che abitano alla Banca centrale di Francoforte, i masochisti che non comprendono la necessità urgente di foraggiare e promuovere la crescita e il lavoro, stregati come sono, in una logica piccolo-bottegaia, dalle frescacce che loro stessi ci hanno ammannito tutta l'estate sulla grande crisi da debito. Finché gli europei si agitano dentro la crisi con mezzi solo fiscali e stangate dietro stangate» - come quelle che subiranno gli italiani con questa manovra (si tratta di oltre 2.000 euro a famiglia) - «finché la Banca centrale continuerà a comportarsi da ragioniere generale della moneta, applicando una politica della lesina e della castrazione dell'economia reale, punitiva verso il debito e disastrosa per la crescita, l'Europa non uscirà da una spirale

più rigorosa, vale per la Grecia ma non vale per la Spagna e per l'Italia che hanno situazioni debitorie e patrimoniali di deficit sostenibili. La differenza è che alcuni Paesi, come la Gran Bretagna, hanno una moneta e possono finanziare il loro debito mentre noi, stando nell'euro, non

L'incentivazione dello sviluppo e la creazione di lavoro sono i veri problemi delle economie europee, come dimostrano i drastici deprezzamenti di borsa nel settore manifatturiero e i dati - quelli sì allarmanti - della produzione in luglio.

perché anche la Corte dei conti ribadisce che la riduzione dell'indebitamento realizzata lo scorso anno non comporta il ritorno ad una gestione ordinaria del bilancio pubblico, perché è ancora incompleto il riassorbimento degli effetti associabili alla crisi dell'economia e vi è l'esigenza addizionale di assicurare, nella prospettiva di medio termine, la coerenza tra i programmi delineati nel DEF e gli impegni, peraltro ancora non formalmente assunti, derivanti dalle nuove regole di *governance* europea. Noi, signor Presidente, abbiamo sempre fatto proposte serie, anche nell'ultima manovra. Avevamo proposto di far pagare quelli che non hanno mai pagato, da sconosciuti al fisco;

dichiarano un reddito oltre il milione di euro, ossia lo 0,01 per cento dei E con chi si accanisce questo Governo? Con i soliti noti, con quelli che continuano a pagare perché hanno la ritenuta alla fonte e che non possono evadere.

invece si è timidi rispetto agli evasori fiscali, che sono stati premiati anche dal Ministro dell'economia, che hanno rimpatriato 105 miliardi di euro. Una patrimoniale del 20 per cento su questi signori avrebbe fatto rientrare 21 miliardi di euro e avrebbe dato un segnale ai contribuenti onesti. Si è scelta un'altra strada. Noi ce ne rammarichiamo, ma bisogna cambiare paradigma. Solo in questo modo il Paese si potrà salvare, e noi facciamo il tifo, anche se i CDS, ossia i *credit default swaps*, che assicurano il rischio Paese, questa mattina sono andati alle stelle

sono state già fatte dal senatore Giaretta, e comunque si è svolto un dibattito abbastanza ampio in Commissione bilancio sul sul rendiconto e sull'assestamento. Pertanto, svolgerò solo alcune sottolineature per rendere più evidenti all'Aula alcuni contenuti dei documenti contabili di grande rilevanza che devono porci, soprattutto in questa fase così complicata per la vita del Paese e per la finanza pubblica, seri interrogativi, più di quanto sia avvenuto negli anni precedenti. L'esame parlamentare del rendiconto ‑ inizio dal rendiconto ‑ è o dovrebbe essere un atto particolarmente rilevante nel corretto funzionamento di una democrazia parlamentare. È il controllo che il Parlamento opera *ex post*, a consuntivo sulla gestione affidata al Governo rispetto a quanto era contenuto nel bilancio di previsione. Quindi, vengono in discussione le valutazioni sui risultati della gestione della gestione della finanza pubblica, sulla attendibilità delle previsioni che erano state fatte con il bilancio di previsione, sull'apprezzamento del definitivo accertamento dei saldi che vengono con questo atto legislativo,

per il rendiconto, oltre le valutazioni politiche sulla gestione della finanza pubblica, è il grado di affidabilità, delle valutazioni effettuate. Ora - come è noto ai colleghi - sul rendiconto la Corte dei conti è

come il momento di congiunzione tra il potere di controllo e la funzione giurisdizionale della Corte dei conti, quindi un qualcosa che unisce le due funzioni fondamentali della Corte dei conti. Quest'anno, signor Presidente, signori del Governo e onorevoli colleghi, il giudizio della Corte dei conti è particolarmente severo. In tutti gli anni precedenti era stato un giudizio critico, a volte molto critico, lo è nei termini che vengono riassunti nel giudizio medesimo e che io voglio espressamente richiamare. Dice la Corte dei conti che il bilancio di competenza, giuridico, sarebbe in parte non trascurabile - sottolineo in parte e non rispecchia in modo fedele l'effettiva realtà contabile, che peraltro, allo stato, è impossibile accertare. In sostanza, la Corte dei conti sostiene che le valutazioni contenute nel rendiconto, che dovrebbero essere basate

di inaffidabilità nella valutazione conclusiva dei conti dello Stato è una cifra accettabile: faccio notare al riguardo che l'8 del bilancio dello Stato, che ammonta ad oltre 800 miliardi, signor Presidente, costituisce una cifra che si aggira intorno ai 65 miliardi di euro. Dunque, la Corte dei conti dice che per 65 miliardi di euro il rendiconto non è affidabile, e non è una cosa di poco conto. Peraltro, specifica anche dove non è affidabile con una elencazione di riscontri, di valutazioni, che non richiamo per ragioni di brevità, se non per due voci. La prima è quella dei residui attivi e passivi, che crescono in modo abnorme; residui che già l'anno scorso avevano subito un'impennata notevolissima, sottolineata dalla stessa Corte

con un incremento rispetto al dato dell'anno scorso di oltre il 12 per cento. Non si comprende qual è la natura di un accrescimento tanto rilevante.

che per una delle macrovoci che compongono il lato delle entrate del bilancio dello Stato ci si sbagli in sede di previsione in misura tanto macroscopica? Questo dato peraltro è una costante negli ultimi 2-3 anni. L'anno scorso si verificò uno abbiamo formulato questa domanda al Governo, che ci ha dato una risposta che, se possibile, aggrava il sospetto di inaffidabilità di dette valutazioni

perché - se non ho capito male - vengono contabilizzate, correttamente da quel lato, dalle agenzie delle entrate le sanzioni e gli oneri accessori sugli accertamenti tributari, che per loro natura sono destinati ad essere oggetto di contenzioso e quindi a rimanere non riscuotibili per lunghi anni. Il che significa che il consuntivo, il rendiconto dello Stato, si basa su una previsione conclusiva, non più preventiva, di un'entrata, quella per sanzioni ed oneri accessori derivanti dagli accertamenti tributari, che non si sa se (e sottolineo se) e quando verranno riscossi. Ecco perché quest'anno, signor Presidente, il giudizio severo Corte dei conti ha un'incidenza molto particolare. o in un consiglio comunale o in un consiglio provinciale e i revisori dei conti avessero formulato rilievi di tale pesantezza, noi avremmo senz'altro il dovere di rispedire al mittente, all'organo esecutivo, questi documenti contabili: non c'è alcun dubbio su questo. Altrimenti approveremmo un bilancio inattendibile, e i bilanci inattendibili sono per loro natura falsi, cioè non veritieri. Siccome siamo in sede in sede legislativa, non corriamo questo rischio, ma ne corriamo uno ben più rilevante, quello cioè di consegnare al prossimo i risultati del rendiconto costituiscono la base per costruire le previsioni del prossimo anno e quindi influiscono sul futuro e non sono soltanto rilevanti per il passato, rilevanti per il passato, dati non attendibili, nella costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, con tutto ciò che ne consegue. Infine, signor Presidente, una considerazione sul bilancio di assestamento. Il bilancio di assestamento, com'è noto, aggiorna le previsioni iniziali del bilancio. Il bilancio iniziale iniziale è basato sul quadro macroeconomico incorporato nella Decisione di finanza pubblica per il triennio 2011-2013. Questo documento, il DFP, fu approvato nel settembre 2010, quindi l'aggiornamento che noi facciamo è su quel dato del dicembre 2010. Noi sappiamo che quest'anno abbiamo approvato il DEF, nella sua prima versione, anticipandolo rispetto alle scadenze tradizionali, che erano quelle di luglio di ogni anno, a seguito della riforma della *governance* economica europea. le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica che erano contenute nel DFP, nel nel documento programmatico del 2010, sono preistoria rispetto agli attuali dati di finanza pubblica. I dati contenuti nel DEF dell'aprile 2011 sono ampiamente superati. Non solo, ma noi tutti sappiamo benissimo che negli ultimi due mesi sono state fatte due manovre di una entità notevolissima. Di tutto questo, dell'evoluzione così marcata dei conti pubblici non c'è traccia nel bilancio di assestamento. caso, noi in Commissione abbiamo sollevato questo problema, abbiamo chiesto al Governo se non fosse il caso di presentare, da parte del Governo, ovviamente, che ha gli strumenti per farlo, un emendamento all'assestamento del bilancio per incorporarvi gli effetti sull'anno corrente, che ci sono e sono rilevanti, delle due manovre di luglio e di agosto. Naturalmente il Governo è rimasto silenzioso, come spesso accade. Non si tratta quindi, signor Presidente, di un di un bilancio di assestamento, perché questo bilancio, che dovrebbe assestare le previsioni acclarate, non assesta proprio un bel niente. La realtà ha assestato molto di più di quanto è contenuto in un documento che siamo chiamati ad approvare, ma che è superato dall'evoluzione rapida dei dati di finanza pubblica a cui assistiamo in questi mesi e in queste settimane. Queste sono alcune delle ragioni (altre sono state già esposte, e altre ancora saranno esposte nella dichiarazione di voto

Grazie, il Parlamento, titolare del potere autorizzativo della spesa, conseguente al prelievo fiscale con cui viene finanziata, accerta la corrispondenza

l'elaborazione del rendiconto e dell'assestamento, che ne rappresenta la naturale conseguenza, traducendo in termini di rettifiche al bilancio le risultanze del rendiconto medesimo, avvenga nel momento in cui la condizione di emergenza della situazione economica generale e specifica del nostro Paese ha già determinato un'ulteriore variazione dell'orizzonte in cui tali atti vengono a collocarsi. Infatti, la predisposizione di rendiconto e assestamento risale allo scorso giugno, ben prima che le turbolenze registrate sullo scenario mondiale e l'attacco speculativo al sistema finanziario italiano, avessero prodotto i loro primi effetti, anche normativi, con due imponenti e profonde manovre, con effetti notevolissimi già sulle risultanze del 2011. Occorre dunque valutare i documenti oggi sottoposti all'esame dell'Aula con la necessaria ponderazione, in considerazione del fatto che le manovre finanziarie operate dal Governo hanno sostanzialmente modificato alcuni fondamenti della finanza pubblica, in ciò determinando anche variazioni di cui non si potrà non tener conto già nell'esercizio in corso, e che emergeranno in tutta la loro rilevante dimensione nel consuntivo 2011 e in parte già con emendamenti sull'assestamento oggi al voto. Uno degli elementi più importanti che emerge dal rendiconto è che già nel 2010, a prescindere dagli effetti delle recenti manovre, i conti dello Stato italiano fanno registrare una inversione di tendenza rispetto all'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Ciò è un dato incoraggiante che riporta il Paese su un cammino virtuoso di riduzione del *deficit* in prospettiva del debito, un cammino che era stato seguito con decisione a partire dal 2006 in avanti, per toccare il livello minimo del *deficit* nel 2008 e che ha subito una brusca interruzione a causa degli oneri che lo Stato ha dovuto accollarsi sia in termini di maggiori spese che di minori entrate, come effetto della recessione nell'ultimo triennio. Peraltro, la condizione di alto indebitamento dell'Italia non ha permesso, come è noto, la predisposizione di misure così massicce come quelle poste in atto da altri Stati europei e dagli Stati Uniti d'America, ma gli effetti - soprattutto in ragione della riduzione delle entrate fiscali - sono comunque stati rilevanti sui conti pubblici. Il miglior risultato del 2010 rispetto al 2009 è da ascrivere sia a una pur lieve, ma comunque politicamente, significativa, riduzione della spesa corrente

tutte le voci di spesa, ad eccezione delle voci di trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, che quindi hanno anche un effetto dovuto al processo di

di trasferimenti correnti all'estero e di trasferimenti correnti alle imprese, tutte le altre voci sono in riduzione, come purtroppo è in riduzione anche la voce investimenti. E questa è certamente una una negatività, ma non poteva essere altrimenti. Prendendo invece in considerazione il lato delle entrate, si deve segnalare un lievissimo incremento, pari allo 0,1 cento: ricordiamoci però che l'anno nero, il 2009, aveva avuto un decremento molto maggiore, pari al triplo. Altre non meno significative considerazioni si ricavano dal confronto tra le previsioni di bilancio e i dati definitivi del rendiconto, determinati nel corso della gestione, con accertamenti che ammontano a 505 miliardi, a fronte dei 507 miliardi e spese finali attestate a 527 miliardi, in riduzione di oltre 13 miliardi rispetto al 2009. Questo è un altro dato importante e significativo.

esame da cui emerge l'importanza delle relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, concretizzata in trasferimenti al sistema degli enti locali, per un importo corrispondente al 26 per cento della spesa. Tale incidenza - come ho già accennato in precedenza - è cresciuta di due punti percentuali rispetto al 2009. A seguire - vorrei ricordarlo - si deve rilevare la significatività della spesa previdenziale, che assorbe circa il 17 per cento totale (elemento di dibattito politico sulle varie manovre), mentre alle politiche economiche, finanziarie e di bilancio va circa il 14 per cento e all'istruzione il 9,6 cento. Distinguendo invece tra spesa corrente e spesa d'investimento, bisogna rimarcare come il 90 per cento del totale vada alla spesa corrente, e alla spesa per investimento meno del 10 per cento, quindi con una riduzione anche rispetto ai periodi precedenti. precedenti. Dal complesso dei provvedimenti, rendiconto e assestamento, oggi all'esame dell'Assemblea, seppure con la precisazione iniziale che entrambi i documenti sono stati redatti precedentemente alle ulteriori evoluzioni del quadro economico, registrate nei mesi di luglio e di agosto, e alle conseguenti manovre correttive messe in atto, emerge dunque, scontando un difficile frangente come quello che indubbiamente è stato l'anno 2009, la capacità dell'amministrazione pubblica di esercitare uno stretto controllo degli elementi determinanti del bilancio sia sul lato delle entrate che delle spese, con un miglioramento generale delle condizioni della finanza pubblica, tale da reinserire il Paese su un cammino di recupero di una maggiore stabilità finanziaria che la crisi economica mondiale aveva messo seriamente a rischio e mette ancora a rischio in questo frangente.

continuiamo ad assicurare le condizioni di lavoro, perché non è possibile andare avanti con questo brusìo che sommerge. volevo in particolare riprendere, tra i tanti interventi, comunque interessanti, che sono stati svolti, quello del collega Giaretta, perché condivido pienamente l'impostazione

Mi piace che abbia ricordato questa contrazione della spesa corrente: quindi, sui dati che anch'io ho evidenziato emerge una sempre più incisiva azione del Governo e del Parlamento sul controllo dei conti. Queste ultime manovre che abbiamo adottato proprio negli ultimi mesi testimoniano ancora questa particolare attenzione alla stabilità finanziaria, che poi è il presupposto anche per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese. Non comprendo invece il collegamento fatto alla questione che riguarda la scuola. Ci sono molte risorse male impegnate e male allocate in alcune realtà del nostro Paese, non è detto che i tagli vadano sempre a eliminare servizi: i tagli puntano ad eliminare gli sprechi, bisogna riallocare e usare meglio le risorse. In tante realtà del Paese, anche in quella in cui vivo, nel mio Veneto, queste drammaticità che sono state evidenziate per quanto riguarda la scuola non esistono, il che vuol dire che ci possono

Signor Presidente, svolgerò una brevissima replica. Il dibattito si è concentrato su aspetti di carattere generale legati ai problemi attuali dell'economia e della finanza. Su molte questioni il Governo, che ringrazio in questa sede, ha dato già risposte credo esaurienti in Commissione, di cui abbiamo parlato anche nella relazione iniziale.

questo passaggio, sia nel rendiconto che nell'assestamento esistano numeri che ci fanno affermare il contrario, cioè la tenuta e la credibilità degli strumenti messi in campo dal Governo in questi anni, pur in condizioni

da sottolineare, e ritorniamo ad avere un notevole avanzo primario ed è questo che ci consente di intaccare o quantomeno di non aumentare per il futuro il debito pubblico. Per quanto riguarda invece le osservazioni avanzate nel dibattito dal senatore Legnini,

sia aumentato il monte residui. Per quanto riguarda il discorso delle entrate extratributarie, il Governo ha fornito una risposta esauriente in Commissione: è dovuto all'enorme ammontare dei contenziosi e delle sanzioni che fanno capo all'Agenzia delle entrate. In merito, è chiaro che si registra una volatilità delle previsioni a inizio anno, ma questo dato contenuto nel rendiconto, e quindi nell'assestamento, è secondo noi più che affidabile.

si è rivolto alle amministrazioni fornendo precise indicazioni, sia per la spesa sia per le entrate. Devo sottolineare, innanzitutto, per la spesa, che l'attività è stata considerata dalle amministrazioni proponenti in funzione delle unità di voto parlamentare costituita - per la prima volta nel corrente anno finanziario - dai programmi, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti dalle missioni. Le proposte di assestamento formulate dalle amministrazioni sono state sottoposte, come di consueto, ad attenta, scrupolosa e rigorosa revisione, comunque strettamente in linea con le indicazioni di cui alla suddetta circolare. Si è proceduto Si è proceduto accogliendo soltanto le proposte conseguenti a imprescindibili esigenze di spesa connesse direttamente a disposizioni legislative, la cui puntuale definizione non può che essere riferita al provvedimento di assestamento, e quelle relative a mere regolazioni contabili e debitorie non aventi impatto sui conti pubblici. Le integrazioni registrate con il presente provvedimento sono complessivamente compatibili con i tendenziali a legislazione vigente per l'anno 2011 contenuti nel Documento di economia e finanza presentato lo scorso mese di aprile al Parlamento. alle integrazioni proposte per gli stanziamenti di spese finali di competenza, esse risultano complessivamente compensate, anche per quanto riguarda il saldo netto da finanziare. Infatti, il provvedimento di assestamento per l'anno 2011 registra riduzioni di spesa per interessi sui titoli del debito pubblico, sui prestiti vari ed altre operazioni finanziarie, per circa 6,1 miliardi di euro, relativi a: per 2 miliardi, alla dinamica degli interessi sui BTP; per 2,5 miliardi, alla dinamica degli interessi sui BOT; per 900 milioni, agli interessi sui CCT e CTZ; per 700 milioni, agli interessi sui prestiti esteri dovuti a minori emissioni. Detta minore spesa, peraltro, è già scontata nei tendenziali a legislazione vigente contenuti nel Documento di economia e finanza. Si registrano, peraltro, minori spese anche riguardo alle somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'Unione europea, a titolo di risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo e sull'imposta sul valore aggiunto. La riduzione proposta, per 600 milioni di euro, è motivata dal previsto conguaglio positivo a favore dell'Italia derivante da eccedenze del bilancio comunitario riferite all'esercizio 2010. Per le entrate, il provvedimento di assestamento registra aumenti delle entrate tributarie pari, nel complesso, ad euro 5.587,5 milioni, 5.587,5 milioni, al lordo dei rimborsi IVA, finalizzati ad allineare le previsioni del bilancio 2011 sia al quadro macroeconomico per l'anno corrente, assunto a base per l'elaborazione delle stime per l'anno 2011 contenute sempre nel citato Documento di economia e finanza, sia ai risultati registrati nello scorso esercizio In ordine al rimborso di prestiti, la riduzione di 16 miliardi di euro viene proposta: per 10 miliardi di euro, a seguito delle minori esigenze di effettuare concambi tra i nuovi CCT ed i vecchi, nonché, per 6 miliardi di euro, per minori rimborsi di prestiti esteri ascrivibili al minor uso, rispetto a quanto previsto, dello strumento delle *commercial Nel provvedimento risultano, inoltre, ricomprese talune integrazioni delle dotazioni di cassa resesi necessarie a seguito dei maggiori residui passivi accertati in sede di chiusura del rendiconto 2010, in gran parte corrispondenti a crediti vantati nei confronti delle amministrazioni, per circa 10 miliardi di euro, di cui 6 miliardi per consentire il pagamento di residui in favore degli enti previdenziali. Per l'importo di 2 miliardi è stato altresì integrato l'apposito fondo cassa. Anche dette integrazioni risultano compatibili con il livello programmato di fabbisogno indicato nel richiamato documento programmatico. nel complesso, risultano quindi effetti positivi sul saldo netto da finanziare, in termini di competenza, per 5 miliardi di euro al lordo degli interessi, restando sostanzialmente neutrali gli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno statale. Devo solo delle precisazioni ad alcuni dei senatori intervenuti in questo dibattito. Con grande piacere, il Ministero dell'economia ha accolto

cui stiamo discutendo, non solo sono affidabili, ma danno anche garanzie e certezze sul futuro del bilancio dello Stato e sulle prossime decisioni che andremo ad assumere. si potrà fare di più, ma in Commissione le risposte sono state date tutte, caro senatore Legnini, e nessuno si è mai rifiutato o è stato reticente di fronte alle richieste che lei ha fatto. Il Governo ha risposto in tutte le occasioni. Lei arbitrariamente vuole offendere il Governo, ma noi non intendiamo assolutamente seguirla su questo terreno. *(Applausi dal

ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, una volta conclusa la votazione degli articoli del rendiconto, si passerà direttamente all'esame degli articoli dell'assestamento. Seguiranno poi le dichiarazioni di voto congiunte e avranno quindi luogo le due votazioni con il sistema elettronico.

di rispettare la legge di contabilità dello Stato, che, all'articolo 17, prevede in modo molto chiaro che alla legge di stabilità siano allegati i documenti programmatici aggiornati

c'è una legge dello Stato che non valuta la possibilità che il Governo dia un aggiornamento programmatico di come intende impiegare le risorse del FAS, ma vincola, obbliga non possiamo accettare che il Governo ci dica, tradotto in un linguaggio semplice, che non rispetterà l'articolo 17 della legge di contabilità dello Stato e che valuterà la possibilità, l'opportunità, di dire o non dire al Parlamento cosa

nel corso dell'audizione svoltasi presso le Commissioni esteri di Camera e Senato, il ministro Frattini, nell'illustrare una serie di interventi che l'Italia intende portare avanti in Libia, nella nuova Libia, ha detto testualmente: «Voglio dire al Parlamento che per attuare queste priorità intendiamo destinare quei fondi che con un impegno del Parlamento stesso e del Ministero dell'economia e delle finanze dovranno essere ripristinati. Si tratta di 8 milioni in assestamento e di ulteriori 8 milioni con la legge di stabilità che, come ricorderete, furono decurtati dal decreto missioni e che il Parlamento e il Ministero dell'economia ripristineranno.

la nuova Libia ed il fatto che il Governo, per bocca del Ministro degli esteri, conta sul ripristino di fondi che erano stati tagliati nel decreto missioni. vi era un accordo *bipartisan*, un accordo tra noi, tra maggioranza e opposizione perché venissero ripristinati. Tale accordo è stato assunto nella solennità di questa Aula a nome del Governo dal sottosegretario Mantica e poi è stato riversato in un ordine del giorno condiviso

in Commissione bilancio il Sottosegretario, a nome del Governo, ha detto che i soldi non ci sono. Mi permetto solo di ricordare un'ultima cosa, perché vorrei che restasse agli atti. Il ripristino di questo taglio era stato chiesto da noi con maggiore forza proprio in considerazione del fatto che, invece, nel decreto missioni il Governo questi stessi 16 milioni di euro li aveva trovati per finanziare l'operazione con cui regalava alcune motovedette italiane a Panama.

noi metterci per traverso su questa vicenda, a prescindere dagli aspetti legali che sono all'attenzione della magistratura. Ma la domanda che abbiamo posto allora e che ripetiamo oggi è: perché finanziare questa operazione con i fondi della cooperazione? Francamente troviamo che ciò sia assolutamente sbagliato.

poc'anzi espresse in modo articolato del senatore Ferrara. I documenti che abbiamo discusso rappresentano certamente l'immagine di un Paese in difficoltà, ma anche l'immagine di un Governo che ha fatto in modo che le difficoltà fossero contenute o comunque rientrassero all'interno dei parametri stabiliti di volta in volta dall'Unione europea. Vi sono molti interventi ancora da compiere e molte iniziative da realizzare. Bisogna soprattutto prevedere interventi specifici che riguardano il rilancio dell'economia. Bisogna pensare a tutte quelle imprese che in questo momento vivono condizioni di disagio perché non sono state ancora pagate per le prestazioni o per i beni forniti alle pubbliche amministrazioni. È necessario che si sblocchi questo circolo vizioso, che

sociale ed infrastrutturale che mostra il nostro Paese e che gli impedisce di presentarsi dinanzi all'Unione europea con un piano di sviluppo realmente efficace, in grado di affrontare la crisi globale con maggiore determinazione.

come se fosse un documento di pura tecnica di bilancio. In realtà, non è così, come ha messo in risalto anche la Corte dei conti nel momento in cui ha evidenziato la necessità di considerare l'assestamento di bilancio un provvedimento di fondamentale importanza soprattutto nei termini della flessibilità dei conti. Crediamo che di questo documento si debba dare anche una chiave di lettura politica per comprendere la condizione nella quale sta operando il Parlamento in questi mesi. Signor Sottosegretario, lei ricorderà che a maggio la maggioranza ha approvato il decreto-legge sullo sviluppo che di sviluppo, poi, aveva solo il nome. venne a riferire alle Commissioni riunite che avrebbe provveduto soltanto con un'operazione di manutenzione ordinaria. Poco dopo, nel mese di luglio, arrivò una mazzata di manovra sugli italiani di circa 40 miliardi di euro e ancora dopo, nel mese di agosto, un'altra manovra di oltre 48 miliardi di euro. In questi giorni, mentre l'Europa da più parti ci sta chiedendo di con misure aggiuntive, il Ministro dell'economia ha dichiarato pubblicamente che farà soltanto un "tagliando". signor Sottosegretario, qualcuno dovrà pur dire al Ministro dell'economia, tra manutenzioni ordinarie e tagliandi, di chiudere questa officina meccanica che sta creando

6 miliardi e 900 milioni di euro: si tratta delle mancate erogazioni dello Stato alle Regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione IVA, e dovrebbero consistere nelle risorse che le aziende sanitarie del Paese dovrebbero usare, a loro volta, per pagare i beni e i servizi e per pagare le piccole imprese. questa maggioranza e questo Governo si strappino le vesti per vedere come accelerare il pagamento alle piccole e medie imprese del nostro Paese se poi lasciamo questo incremento di residui passivi fotografati nell'assestamento di bilancio. esame è un provvedimento, signor Sottosegretario, che nasce già vecchio. Un provvedimento che è fuori dal tempo e fuori dallo spazio fotografa una riduzione degli interessi per il servizio del debito pari a circa 6 miliardi di euro.

il quale vengono usate le risorse del FAS, mediante variazioni compensative per atto amministrativo e quindi non attraverso un impiego specifico di capitoli specifici,

al momento decisivo in cui presenterà la legge di bilancio dello Stato, perché in quel momento l'articolo 17 - come le dicevo, signor Sottosegretario - diventa poi avanti anche sulla questione dell'aumento delle spese, perché in questa sede è stato detto che i conti tornano. Non è vero, perché in termini di cassa c'è un peggioramento dei conti pubblici e un incremento della spesa corrente primaria al netto degli interessi per la bellezza di 9 miliardi di euro. Allora diventa più che mai attuale il contenuto dell'emendamento che i colleghi del Partito Democratico hanno presentato in occasione della manovra di agosto che abbiamo votato,

specifico da introdurre nell'ultima manovra, perché è già legge dello Stato. Si tratta del decreto-legge n. 98 che è stato convertito in legge e che, all'articolo 9, stabilisce che il Ministro dell'economia deve indicare al suo Ministero un atto di indirizzo per avviare il ciclo della revisione della spesa. Al mese di settembre stiamo ancora aspettando questo atto di indirizzo. Allora, sulla base di queste quattro criticità, signor Sottosegretario, si rende conto che non abbiamo alcun elemento per poter votare questo disegno di legge di assestamento del bilancio, soprattutto se lo si vede nel contesto economico e sociale nel quale viviamo. Mi avvio alla conclusione leggendo un commento, un giudizio molto importante che è stato dato da un quotidiano molto seguito a livello internazionale e molto apprezzato anche a livello nazionale, il quale dà una fotografia dello stato che vive il nostro Paese. Leggo testualmente, signor Sottosegretario: «Il fallimento dello Stato non è mai stato così vicino. Anche ieri siamo stati salvati dalla Banca centrale europea. Fortunatamente da Berlino hanno lasciato comperare i nostri soldi. Basta questo per stare tranquilli? No. Da Bruxelles hanno fatto capire che il conto fatto sulle entrate della manovra in corso di approvazione non va in copertura del debito come auspicato. Si renderà necessaria una manovra aggiuntiva. Quello che entrerà non basta. Allora giù la maschera. Il tempo delle finzioni è finito». Signor Sottosegretario, queste parole non sono riportate nell'editoriale del «New York Times», del «The Daily Economist» che ce l'ha con il presidente Berlusconi o del «The Washington Post». Sono le parole le parole pubblicate ieri, soltanto ieri, nell'editoriale del quotidiano «La Padania», il giornale di partito del vostro maggiore alleato. Signor Sottosegretario, riferisca agli altri componenti del Governo di gettare giù la maschera e di smetterla con le finzioni. Il Paese non può più attendere. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, l'esame del rendiconto dovrebbe servire ad esaminare, sui dati veri o quantomeno sui dati *ex post*, l'andamento dei fondamentali della finanza pubblica e servire quindi, fondamentalmente, a due cose: post* gli orientamenti a suo tempo stabiliti con i bilanci preventivi - in questo caso, con il bilancio del 2010 - e le varie misure finanziarie assunte, valutare gli scostamenti e interpretarne le ragioni, valutare lo stato delle finanze che si è conseguentemente determinato, e in secondo luogo servire da base per adeguare il bilancio il bilancio dell'anno immediatamente successivo. Questo avviene con l'assestamento, che è infatti il provvedimento esaminato parallelamente al rendiconto. La prima osservazione da fare, svolta nel corso del dibattito odierno, è che purtroppo sulla veridicità e attendibilità di questi dati il giudizio della Corte dei conti è molto pesante e getta una luce piuttosto fosca su quanto abbiamo cercato di esaminare. Non di meno, se vogliamo fare qualche osservazione da cui discendono le nostre valutazioni e il nostro orientamento di voto in ordine alle ragioni degli scostamenti, alla valutazione dello stato reale dei conti pubblici che ne consegue e alle proposte per l'assestamento del 2011,

quali a causa della crisi economica i conti avevano segnato un brusco e deciso peggioramento rispetto agli anni precedenti. Il confronto con il bilancio preventivo del 2010, ed anche con il rendiconto del 2009, evidenzia miglioramenti dovuti ai lavori in corso, che certamente ci sono tuttora con le manovre appena approvate, anche se non incidono sul rendiconto. Con tutto ciò l'entità delle variazioni, anche se qualche volta è significativa, appare modesta e insufficiente rispetto all'enormità del lavoro da fare. Sembra si possa dare conto di tagli e di sforzi ma non certo di una svolta. In realtà, è proprio di una svolta che vi sarebbe bisogno anche se questi indicatori del rendiconto non sono quelli che formano i parametri di Maastricht, basati su un altro aggregato di tutte le amministrazioni pubbliche, tuttavia l'influenzano moltissimo. Questi parametri, per il 2010, sono mediamente i secondi peggiori del decennio dopo quelli del 2009. Lo è il parametro dell'indebitamento netto rispetto al PIL; lo è quello del saldo primario rispetto al PIL, tornato negativo proprio nel 2009 dopo essere stato

che questi indicatori non nascono solo dal rendiconto ma in gran parte da esso, ma siamo anche consapevoli che questi indicatori si sono molto aggravati, soprattutto per effetto della caduta del denominatore, cioè del PIL. Tuttavia, è evidente che di fronte a questi dati è proprio la svolta che non c'è stata ciò che sembra emergere dal rendiconto in esame. Venendo proprio ai dati del rendiconto, si evidenzia un certo miglioramento degli andamenti gestionali, anche se non privo di qualche ombra. Il saldo netto da finanziare è sceso, come è stato correttamente rilevato, e così il ricorso al mercato finanziario, anche in modo consistente. Tuttavia le dinamiche di cassa attestano complessivamente una gestione in peggioramento, sia pure leggero. Il saldo di competenza delle partite finali resta negativo, anche se migliora un po' sul 2009, ma dal punto di vista delle entrate si registra una riduzione del gettito tributario ed una riduzione delle entrate extratributarie. Il saldo netto da finanziare - lo abbiamo detto - è diminuito, ma al tempo stesso c'è un incremento, ancorché lieve, del quindi un andamento in chiaroscuro con qualche miglioramento, ma certamente non una svolta, come conferma anche la torta che illustra l'andamento delle spese divise per missione, secondo le nuove regole della legge di contabilità contabilità pubblica, da cui emerge che il debito pubblico continua a fare la parte del leone (e questa è una grande palla al piede) e, fatto cento l'insieme degli altri utilizzi, i trasferimenti agli enti locali pesano per il 26 per cento, le politiche previdenziali per il 17 per cento, l'istruzione scolastica per il 10, essendo costituita

per la loro valutazione, chiama in causa il tema dell'affidabilità degli accertamenti e, quindi, ha conseguenze sulla qualità e attendibilità dei dati contabili. C'é poi il tema del patrimonio, il cui valore peggiora, e non dimentichiamo che per la legge di contabilità esiste l'obbligo di individuare i beni suscettibili di utilizzazione economica, anche per valutare l'analisi economica della gestione patrimoniale. Le informazioni al riguardo, tuttora incomplete, devono sovrintendere al processo di federalismo E poi c'è, molto grave, sul fronte delle spese, il problema delle eccedenze sulle previsioni definitive di competenza e delle spese effettuate in mancanza di stanziamenti in bilancio, registrate nel consuntivo come eccedenze: la Corte dei conti eccepisce che questo modo di fare non è regolare e chiaramente si tratta di soluzioni sbagliate non solo nella

previsioni in termini di cassa determina nel 2011 un peggioramento dei saldi. Quindi ci sono effetti divergenti del disegno di legge sul saldo di cassa rispetto a quanto si registra sul versante della competenza. La differenza è riconducibile proprio al lato della spesa, in particolare della spesa corrente (che aumenta di 9,4 sono poi alcuni problemi aperti o risolti negativamente che sono stati trattati in questo dibattito, quello dell'utilizzo del FAS, su cui non torno, o quello dei residui passivi che ritorna anche in questa sede e per questi motivi appare insufficiente e inadeguato l'insieme delle indicazioni di cui alla proposta del disegno di legge di assestamento. Alcuni punti si possono ricordare brevemente, ma ce n'é uno su cui mi premeva attirare l'attenzione una delle indicazioni della legge che andiamo a votare fra poco: il Ministro dell'economia e delle finanze sarà autorizzato a variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli dei versamenti all'Unione europea per l'IVA e per i dazi. Questa è una cosa piuttosto curiosa e mi sarebbe piaciuto capire, dall'esame del testo di legge (e non è possibile), quali sono le motivazioni per questo. In conclusione, pur a fronte di miglioramenti apprezzabili nei conti della pubblica amministrazione, non solo non vi è il segnale di una svolta, ma vi sono al contrario molti motivi di preoccupazione e puntuali rilievi della Corte dei conti che rimangono senza risposta o, peggio, rimangono con una risposta assolutamente negativa.

Posto che non si può pensare di risolvere questo problema solo con la crescita, possiamo pensare di agire con un recupero netto di risorse, quindi abbattendo il debito. Ebbene, dovremmo abbatterlo di 650 miliardi.

A questo punto che fare? È quello che ci chiediamo noi: che fare? Anche perché si sta cominciando a parlare di doppio euro, e per la Lega Nord è evidente che non esiste neanche la possibilità di non rimanere con l'euro del Nord-Europa. Dobbiamo agire sul lato spese e sul lato entrate. Allora, vogliamo agire sul lato delle spese? Va bene! E' iniziato il processo della *spending review*, il federalismo con i costi *standard*, ma è evidente che qui dobbiamo darci una accelerata, e pure in fretta, perché il 2013 è vicino. Ma poi c'è anche l'altro obiettivo da raggiungere. Allora, rimane da agire sul lato delle entrate. Poiché è impensabile aumentare la pressione fiscale, che è già ai livelli più alti del mondo, bisogna contrastare l'evasione fiscale. Abbiamo sentito da diversi colleghi richiamare il problema annoso dell'evasione fiscale.

la Sicilia 51, la Campania 48. Quindi, dai 148 dell'Emilia-Romagna si arriva ai 50 di media nel Sud. Tradotto in pressione fiscale significa che nella mia Lombardia la pressione fiscale si mangia più del 50 per cento del PIL. In tutto il Sud la pressione fiscale si mangia dal 35 al 38 per Quindi, quando parliamo di evasione fiscale dobbiamo renderci conto di questa enorme ingiustizia esistente nel nostro Paese. andiamo a sommare il dato sul residuo fiscale, cioè la differenza tra quanto una Regione versa e quanto una riceve, abbiamo un altro dato imbarazzante, nettamente correlato a quello della differenza tra consumi e reddito di cui abbiamo detto prima. Ebbene, i miei concittadini lombardi perdono 7.200 euro l'anno. Versano cioè 7.200 euro l'anno in più rispetto a quello che ricevono.

Data la correlazione tra questo dato e quello della differenza tra reddito e consumo, è evidente che abbiamo molto da fare sul contrasto all'evasione fiscale. Però è un contrasto che va fatto, dove l'evasione fiscale ha questi dati assolutamente fuori norma. Ribadiamo e concludiamo dicendo che per la Lega Nord non esiste la possibilità di non rimanere agganciati all'euro forte della Germania e della Francia. Però, possiamo risolvere tale questione solo se risolveremo il problema dell'evasione fiscale fino in fondo.

Su questo atto la Corte dei conti esprime un giudizio molto pesante. Il sottosegretario Gentile se la cava dicendo che il bilancio è affidabile; la Corte dei conti sostiene che in gran parte non lo Allora, se il bilancio è affidabile, non è affidabile la Corte dei conti: mettiamoci d'accordo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Siccome ci sono dei giudici, voi perdete il lume della ragione e cominciate a dire che non è affidabile nemmeno la Corte dei conti. *(Applausi dal Credo che un po' di modestia non guasterebbe. Se i revisori dei conti - come diceva prima il dessero un giudizio come lo dà la Corte dei conti su un bilancio di un Comune, a quel sindaco consiglierei di trovarsi una buona assicurazione. Secondo me, a voi non vi assicura nessuno, con un giudizio del genere della Corte dei conti, perché è un giudizio

È vero che ci sono dei segnali positivi per quello che riguarda il contenimento della spesa. Vorrei però ricordare al Governo che oggi l'ISTAT ha certificato che il debito è arrivato a 1.911 miliardi. Allora, ci saranno pure dei segnali positivi, ma la medicina non è adatta all'ammalato, perché voi state

ha guardato il bilancio, tra residui attivi e residui passivi arriviamo a quasi 300 miliardi, miliardi, quasi alla metà del bilancio, al 40 per cento del bilancio. Ma di cosa stiamo parlando? Residui attivi e residui passivi: vuol dire che la macchina pubblica non funziona.

e il Paese sta entrando in una spirale dove la pubblica amministrazione non paga più. E voi dite che siete contenti? Ma dove esiste una roba del genere? Dovreste fare un atto di modestia e mettere mano alle cose che non funzionano.

aveva impegnato una serie di voci di spesa. Quei 2,4 miliardi saltano fuori per un miliardo da spese che dovrebbero sostenere lo sviluppo, le attività produttive;

questo Paese (si va a tagliare sempre sulle voci che dovrebbero creare crescita e sviluppo) e avete fatto due danni: non avete fatto l'asta per le frequenze e, al tempo stesso, avete tagliato su due voci. Non vi limitate più a un danno per volta: adesso ne fate due per volta, perché non solo non fate non fate l'asta per le frequenze, ma addirittura tagliate i soldi per gli incentivi alle attività produttive e tagliate i soldi per i FAS. Un tale modo di governare è inaccettabile, inattendibile, inaffidabile: chiamatelo come volete.

Signor Presidente, come osservo sempre, in queste occasioni strappare applausi non è difficilissimo *(Applausi come si è dimostrato, peraltro. Ma, nonostante tutto, il compito in questo momento è invece di fare delle analisi il più possibile documentate. Senza allora fare le solite considerazioni di politica generale, che in questi mesi abbiamo più occasioni giustamente per poter fare, è utile analizzare alcune questioni che i due provvedimenti al nostro esame recano. La prima questione è la seguente. Avevo avuto occasione di dire nell'ambito della discussione sull'ultima manovra che questo Governo esegue

come gli altri ne sono infastiditi. fu previsto un introito di 2,4 miliardi di euro per l'asta delle radiofrequenze, per serietà questa norma fu accompagnata da una clausola di salvaguardia la quale affermava: ove mai non si conseguano queste cifre, si effettua un taglio corrispondente della stessa cifra sui Ministeri. Sempre per serietà, agli inizi di quest'anno quella somma di 2,4 miliardi di euro fu accantonata. Si controvertì allora se quella previsione di 2,4 miliardi fosse eccessiva o no: i colleghi della opposizione supponevano che fosse eccessiva, quelli della maggioranza invece erano più ottimisti. Come è andata la questione? Con questa questa manovra, quella di ferragosto, chiamiamola così, la clausola di salvaguardia è stata migliorata, e all'articolo 40 si è detto: quei 2,4 miliardi di tagli di tagli ai Ministeri vengono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, e vediamo poi fra un attimo che cosa succede all'asta delle radiofrequenze. Con questo assestamento sostanzialmente si esegue quella norma, e i 2,4 miliardi vengono destinati integralmente al miglioramento dei saldi. Dunque, quella manovra ha conseguito i suoi effetti in maniera assai assai positiva per la finanza pubblica italiana, ed è giusto dirlo ad alta voce. Ma non si è verificato solo questo a favore della posizione della maggioranza e del Governo: si è anche avuta conferma che avevano ragione ad essere ottimisti.

queste cose, come tutti crediamo, faremmo un bene all'Italia; se si leggessero questi atti sarebbe utile per tutti, anche per quella parola che oggi va tanto di moda, per i «mercati».

alla sostanza delle questioni, perché l'assestamento questo fa e il rendiconto questo fa. Nel FAS, agli inizi dell'anno, per il 2011 (perché solo di quest'anno si tratta, e poi potremo farlo per gli altri anni) c'erano 9,073 miliardi di competenza.

di competenza sul FAS ben 6,5 miliardi. Dunque, facciamo bene a porci il problema che il FAS deve continuare ad essere destinato alle sue finalità specifiche, ma intanto rendiamoci conto che, essendo stato per

con le destinazioni improprie fatte per le somme del FAS, abbiamo ancora oggi, per la sola quota di competenza del bilancio statale (perché - come sapete - abbiamo riprogrammato quella regionale, sempre con la manovra precedente, e anche questo dobbiamo dirlo con orgoglio), 2,5 miliardi di cassa, che potremmo (anzi, dovremmo) spendere entro il 31 dicembre, se non vogliamo che diventi un residuo. Dunque, il problema vero del FAS, da queste cifre, è evidente, sia per competenza che per cassa. E deve esserci uno sforzo di tutto il Parlamento, ma in particolare degli uomini del Mezzogiorno, non soltanto per appostare cifre, ma soprattutto per destinarle e spenderle. Il successo lo avremo quando questa voce, che assume talvolta quasi un carattere mitologico, diventerà voce concreta. Una cifra dal bilancio deve diventare spesa, perché così si sentono gli effetti. Allora, l'auspicio e, più ancora, l'impegno che dobbiamo mettere

non riesce a far spendere è l'insieme straordinario di sovrapposizioni di procedure che insieme, come compito, dovremmo snellire, e con grande rapidità. Mi pare che ciò fotografi l'assestamento. Questi sono i compiti compiti che abbiamo di fronte e questo è lo stato effettivo dell'azione di governo e della maggioranza, che oggi possiamo definire largamente positivo nei confronti di una crisi grave, la più grave che stiamo vivendo a memoria d'uomo, e che dà ancora più conforto all'azione che dobbiamo intraprendere. Certo, ogni azione va sempre migliorata, e certo non disconosco anche le situazioni in cui, con i colleghi dell'opposizione, troviamo significativi momenti d'incontro. Abbiamo mostrato, anche in questa manovra, la capacità di prendere per nome e anche per cognome, le proposte che noi riteniamo di interesse da parte dei colleghi dell'opposizione. Ma, vivaddio, tutti insieme rendiamo al vero Mi pare questo il compito che, con questo assestamento, abbiamo ancora una volta svolto. Per questo motivo, il nostro voto apre una nuova finestra"). Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2803, nel suo complesso.

Tina Richard, una cittadina nigeriana di 28 anni, originaria di Kanu, di religione e famiglia cristiana, rifugiatasi in Italia dopo essere fuggita dal suo Paese all'età di 15 anni a causa dell'assassinio dei suoi genitori da parte di un potente e e facoltoso concittadino che la voleva in sposa ancora ragazzina. Tina, aiutata dal vescovo locale, è venuta in Italia per la prima volta nel 1998. Nel 1999 l'Italia, però, l'ha deportata in Nigeria e possiamo dedurre che cosa è capitato a questa ragazza: torture, stupri, correzioni fisiche e maltrattamenti, perché doveva essere redenta.

bisogna concedere l'asilo: dovrebbe essere un fatto quasi automatico. L'organizzazione umanitaria EveryOne assiste questa ragazza in Italia. Io mi permetto di aggiungere il mio appello a quello di EveryOne e degli avvocati che seguono questa

anch'io mi associo alla richiesta della senatrice Garavaglia, segnalando tra l'altro che la commissione territoriale di Caserta, da quando è stata istituita, peraltro

ricordato poco fa della senatrice Garavaglia sono molti. Rischiamo ancora una volta di violare il diritto internazionale, che invece abbiamo deciso di includere nel nostro ordinamento. **Per un'informativa del Governo Signor Presidente, mercoledì prossimo il Senato terrà una seduta dedicata alla situazione delle carceri nel nostro Paese. Lunedì scorso, insieme ad altri parlamentari e ad una delegazione di rappresentanti sindacali della polizia penitenziaria, sono andato a visitare quello che considero un esempio della cattiva amministrazione penitenziaria del nostro Paese. Si tratta del carcere di Gela, terminato da quasi quattro anni, inaugurato per ben due volte, pronto in ogni sua parte ad essere utilizzato, ma ancora chiuso. Questa situazione costituisce una offesa nei confronti del livello di civiltà del nostro Paese, perché paradossalmente, mentre in Italia sono presenti numerose carceri nuove, ma chiuse, in quelle esistenti e funzionanti i detenuti vivono in condizioni del tutto disumane, come purtroppo sancito persino

possa fornire, tra gli altri, i dati relativi alle carceri esistenti e non utilizzate, con le relative motivazioni, è ovvio, e i dati relativi alla situazione del personale. A quanto pare, infatti, e questo sarebbe molto grave, dato che noi già da più di un anno abbiamo

delle problematiche appena riferite riguarderebbero proprio la scarsa disponibilità di personale, che è certamente sottodimensionato di circa 6.000 unità,